Vorrei ritornare un momento sulle questioni che abbiamo ripetutamente posto in quest'Aula e richiamo l'attenzione soprattutto della Presidenza. Mi riferisco alla questione Visco e al problema delle deleghe. deleghe. Abbiamo richiamato l'attenzione su un fatto, credo, estremamente grave, che io insisto nel riproporre all'attenzione della Presidenza. Accade che siamo in presenza di un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, il n. 53 del 1° giugno 2007, che così recita, tra l'altro: «La delega (comma 3 dell'art. 1 del DPR 7 giugno 2006) è stata avocata dal Ministro dell'economia, Tommaso Padoa-Schioppa». Tutto questo, naturalmente, non ha avuto poi un seguito, come sarebbe stato lecito attendersi, da un

allorquando vengono conferite le deleghe ai Vice ministri, ed è conferita anche quella al vice ministro Visco, viene previsto, al comma 3 «Il potere di direttiva nelle materie delegate viene esercitato dall'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco in coerenza con il generale potere di direttiva intestato al Ministro dell'economia e delle finanze, nel cui ambito, nei confronti della Guardia di finanza, l'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco esercita tutti i poteri delegati ai sensi del comma 2». Ora, noi siamo in una vicenda per così dire oscura, nel senso che andrebbe precisato con un nuovo atto di Governo quali sono le deleghe attribuite al vice ministro Visco e invece tutto questo non c'è. Per tale ragione, signor Presidente, credo sia necessario che il Senato disponga di un nuovo atto di delega preciso, per verificare le responsabilità su tutti gli atti di Governo per come possono essere successivamente imputati. A questo riguardo, signor Presidente, ho presentato una proposta d'inchiesta parlamentare monocamerale, affinché il Senato possa verificare attentamente tutto l'andamento della questione. Senatore Eufemi, non debbo ricordare a lei, che è molto più esperto di me, che il richiamo al Regolamento sostanzialmente si intravedeva con grande difficoltà nelle cose che ha detto. Vorrei dire, sulla vicenda che ha interessato giustamente il Senato ormai da parecchie settimane, che riguarda le questioni collegate alla Guardia di finanza, le vicende del vice ministro Visco, che alle ore 13, quando ci sarà la riunione dei Presidenti dei Gruppi,

*(AN)*. Signor Presidente, nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha sottolineato l'esigenza di un accurato lavoro di prevenzione a fronte del nuovo allarme terrorismo.

noi, infatti, abbiamo appreso dell'esistenza di una circolare trasmessa ai senatori Questori, come atto doveroso che viene assunto in questi casi per richiamare ad una maggiore attenzione e vigilanza; ma sappiamo anche che ciò che è accaduto nel Regno Unito nelle ultime ore fa emergere un tipo di terrorismo che qualcuno ha definito «fai da te» e che richiede un'attività di prevenzione particolarmente analitica e dettagliata. Tutti noi abbiamo inoltre appreso, direttamente o attraverso i *mass media*, dell'enorme carenza di fondi che le forze di polizia ed i Servizi di informazione e sicurezza lamentano a seguito dei tagli della legge finanziaria in vigore, tagli che per i Servizi di sicurezza stanno inducendo al licenziamento di decine e decine di operatori. pertanto indispensabile che il ministro Amato, che proprio in Parlamento - nell'altro ramo - ha denunciato in modo drammatico tale carenza di fondi e di risorse,

è la legge comunitaria 2007, che come di consueto contiene tutte le disposizioni atte ad adeguare la legislazione italiana alle normative comunitarie. La caratteristica della legge comunitaria 2007 è quella di prevedere al suo interno per la prima volta in maniera esplicita l'attuazione di tutte le direttive in scadenza entro i termini di validità della legge.

Il primo elenco, quello cioè di direttive che non passano attraverso il controllo parlamentare, di anno in anno si restringe e dopo l'esame della Commissione è ridotto ad una sola direttiva. La prima parte della legge contiene rispetto agli anni scorsi poche modifiche; quella principale, che costituisce da un certo

Questo dovrebbe consentire di essere puntuali nel recepimento delle direttive comunitarie stesse. La seconda novità è costituita dalla possibilità data al Governo di emanare non solo Testi unici, ma anche codici di materia su argomenti toccati dalle direttive stesse. In sede di discussione in Commissione, questa prima parte ha subito pochissime modifiche; la più rilevante riguarda il tema, già controverso lo scorso anno, della informazione che il Governo deve dare al Parlamento relativamente agli atti che riceve dalla Comunità. Si è cercato di trovare un criterio per cui vi sia l'obbligo di informazione quantomeno per gli atti che sono alla base di disegni di legge di iniziativa governativa o di decreti legislativi. Comunque, questo è un punto delicato su cui forse si dovrà soffermare ancora l'Aula.

norme che cercano di evitare procedimenti di infrazione, a norme correttive di disposizioni precedenti, a direttive recenti, che richiedono o hanno richiesto un intervento più rapido. Spesso si usa la metafora del treno per indicare la legge comunitaria o le leggi analoghe e una metafora può essere utile anche in questo caso: qui si tratta di un treno un po' lento, sul quale, come su tutti i treni lenti, saltano

potenziale difetto dell'articolato che qui presentiamo. della discussione in Commissione si è registrata una novità positiva, nel senso che sono stati man mano presenti, oltre ai rappresentanti del Ministero comunitario, anche rappresentanti dei singoli Dicasteri interessati in quel momento (quindi in materia di agricoltura, di giustizia e di società) e ciò ha consentito un esame abbastanza approfondito. Questa seconda parte della legge comunitaria è quella che ha subìto, anche per quanto detto poco fa, le maggiori modifiche in sede di esame in Commissione. Sono stati eliminati alcuni articoli del disegno originario, in particolare in materia di etichettatura di prodotti agroalimentari, e altri ne sono stati introdotti. Particolarmente significativa è una norma che interviene sul problema del CIP 6 e in sostanza ricalca il contenuto di un analogo disegno di legge presentato dal Governo,

2007 sta nella terza parte, in cui per la prima volta vengono introdotte in legge comunitaria disposizioni in materia di giustizia, cioè decisioni quadro europee. L'inserzione di disposizioni in materia di giustizia nella legge comunitaria è espressamente richiesta dalla legge Buttiglione. In tal senso, il Governo ha compiuto un atto dovuto. Il capo che regola le decisioni quadro si compone di cinque articoli: nel primo sono dettati alcuni criteri generali;

corruzione tra privati, in cui si è seguito un criterio di continuità, nel senso che il Governo ha un presupposto per il reato di corruzione sia la violazione della concorrenza, una riserva che aveva fatto l'Italia nel momento dell'approvazione della decisione comune. Questo criterio è stato mantenuto.

un ampliamento della fattispecie, per allargare la sfera soggettiva dall'ambito delle società a quello di tutte le persone giuridiche ed associazioni private. Le altre decisioni-quadro hanno rilevanza minore, hanno suscitato meno

di sanzioni pecuniarie, di cui comunque si è seguito il modello e lo schema del mandato d'arresto europeo.

che nella discussione in Commissione si è cercato anche di fare piccoli passi nella direzione di rendere un po' più leggibile anche per i cittadini la legge comunitaria per cercare di avvicinare anche l'opinione pubblica comune alle decisioni europee. Per questo, quella che fino ad oggi era la relazione introduttiva della legge verrà in futuro allegata nella legge stessa come una nota addizionale. Questo è un documento assai utile, tra altro l'unico in cui si trova in maniera pubblica tutto l'elenco lunghissimo delle direttive che il Governo si riserva di attuare in sede amministrativa. La Commissione, d'accordo con il Governo, aveva anche proposto una drastica cura dimagrante della legge comunitaria annuale, cercando di trasferire tutta la prima parte nella legge Buttiglione. Però, vi è stato un del tutto condivisibile rilievo della 1a Commissione, che ha fatto notare come una decisione così grave sia un oggetto estraneo alla legge comunitaria stessa. Resta, comunque, in futuro il problema non solo di semplificazione e di snellimento di questa legge, ma anche di un riesame più approfondito, quanto meno su due punti: luogo su tutti i rapporti tra Stato e Regione nell'attuazione delle direttive europee che la legge Buttiglione ha risolto in linea teorica, ma che sul piano pratico crea ancora grossi problemi e che diventa più drammatico con il fatto che oggi le Regioni sono direttamente responsabili delle eventuali sanzioni pecuniarie. Il secondo problema è più generale e deriva dal fatto che l'impianto della legge comunitaria è è nato in un periodo in cui non esisteva ancora in maniera chiara una priorità del diritto comunitario, un'immediata attuazione del diritto comunitario. Quindi, tutta la legge andrebbe probabilmente ripensata alla luce dei nuovi rapporti tra diritto comunitario e diritto statale.

signor Sottosegretario alla giustizia, onorevoli colleghi, in questa nostra discussione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea è certo dominante

spaziare dal controllo all'indirizzo, dal consuntivo a ciò che si dovrà fare.

grande processo di integrazione fra ordinamenti dello Stato che si svolge continuamente, ogni giorno. Un processo segnato da avanzate e anche da resistenze.

Accogliamo quindi con favore gli accordi interistituzionali preannunciati dal Governo per quanto riguarda la fase ascendente e la fase discendente

Occorre cioè che si producano condizioni giuridiche nuove perché questo adeguamento, non certo automatico, avvenga con una rapidità di tempi tale da toglierci dai bassi fondi della classifica, come dicono come dicono i giornalisti sportivi. Con questo non diciamo che il Governo non si sia dato da fare.

disegno di legge comunitaria, il relatore Enriques lo ha detto poco fa, che ha accorciato sensibilmente i tempi di delega: adesso la delega coincide con il termine di scadenza della direttiva ed è solo di 90 giorni, se la direttiva è già scaduta nei tre mesi successivi. Quindi, un sforzo c'è stato, come anche la creazione di una struttura di missione all'interno del Ministero. Tuttavia, tutto ciò non basta. Non basta

l'IPEX, un sistema informatico che ci consente in tempo reale di seguire anche l'attività degli altri Parlamenti. Eppure,

nel fatto che i Governi non sono perfettamente integrati con quanto avviene a Bruxelles. Da questo punto di vista, mi hanno molto impressionato le dichiarazioni iniziali del soggetto

europea. D'altra parte, se valutiamo la fine struttura della strategia di Lisbona e la necessità in cui si trovano i Governi nazionali ogni anno di presentare un progetto nazionale di riforma, vediamo che questo progetto nazionale coincide

di un settore della politica europea, e delle varie politiche nazionali, che corrisponde ad un bisogno intensissimo in Europa: il bisogno di sicurezza.

Il controllo delle frontiere ci porta, poi, inevitabilmente ad un altro aspetto della partecipazione dell'Italia alla politica comunitaria, quello riguardante la

ma ciò che si vuole dire è che questi temi esulano dal classico diritto internazionale per rientrare nel diritto alla sicurezza interna. Ci sono due grandi questioni di vicinato che ci interessano strettamente: i Balcani occidentali e la cosiddetta Unione Mediterranea. Quanto ai Balcani occidentali è sempre più evidente la necessità che il mare Adriatico sia un mare interno all'Unione Europea, un «mare intimo» come ha detto il grande scrittore

ormai l'idea, lanciata dal Presidente della Repubblica francese, di una Unione Mediterranea. Essa è già stata subissata da critiche, «eppur si muove», perché la chiamata di

Certo non siamo soddisfatti di quello che è avvenuto a Bruxelles, ma ci rendiamo conto che è l'inevitabile conseguenza di due *referendum* del no che hanno rappresentato non tanto il ripudio dell'Europa,

attenzione alle reazioni dell'opinione pubblica. Si spiega così sia il ruolo accresciuto assegnato ai parlamenti nazionali di cui dobbiamo prendere atto, sia alcune ambiguità interpretative presenti nel Trattato che, certamente, dovranno essere risolte in seno alla Conferenza

parteciperà, membro tra i membri sotto la Presidenza del lussemburghese Junker, il Presidente della Repubblica francese. È un atto di grande valore simbolico questo. Che cosa vuol dire questo atto? Vuole dire che l'Unione economica

Si sono messi insieme fiori, banane, uova da etichettare con il recepimento di norme sulla giustizia necessiterebbero di una trattazione ben più ampia, in ogni caso separata da un contesto che stride per importanza e peso.

dove la Gran Bretagna - vorrei ricordarlo al Presidente di Commissione - ha ottenuto che le direttive europee sulla giustizia non abbiano il sopravvento sulla giurisprudenza inglese.

la menzione dei cosiddetti accordi quadro tra quelli che possono e devono essere veicolati

che la legge Buttiglione non ha effetti nel nostro ordinamento, determinando un esito assolutamente abnorme. Naturalmente, questa richiesta di non insistenza va collegata

che le decisioni quadro comunitarie in materia di cooperazione giudiziaria, di controllo delle frontiere, possano avere un

che l'integrazione di varie richieste è dovuta a questa necessità imposta dalla legge Buttiglione. È pienamente legittimo, quindi, quel quadro normativo che talvolta può apparire variegato, anche disomogeneo, ma che ha una sua unità sistematica nella esigenza del processo integrativo cui l'Italia deve obbedire, anzi questa volta l'apporto dei singoli rappresentanti dei Ministeri interessati ha consentito non soltanto di dare un contributo in materie specifiche,

tutte ricomprese nel sistema delle decisioni quadro. Dunque, il Governo non soltanto condivide appieno il contenuto della Relazione e la ricca e corposa esposizione

Presidente, la discussione e approvazione della legge comunitaria annuale è un'occasione importante per esaminare i vari aspetti della complessa partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, verificandone lo stato di avanzamento, i benefici, i problemi, le difficoltà e le eventuali conseguenze negative. Al riguardo, opportunamente tale esame parlamentare comprende, da qualche anno, insieme al disegno di legge comunitaria, anche il documento: «Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea» relativo all'anno precedente, presentato dal Ministro in carica per le politiche europee.

Data la complessità e l'ampiezza della gamma delle politiche europee, 300 pagine scarse di relazione sono a mio avviso troppo poche: l'eccessiva sintesi finisce per ridurre la Relazione ad un mero elenco di provvedimenti, privo di incisività e di visione critica, e lo connota in termini di documento burocratico, non politico. Fa specie l'assenza della benché minima contrapposizione o commento negativo, come se qualunque decisione presa a Bruxelles andasse sempre bene all'Italia.

Mancano nella Relazione adeguate valutazioni qualitative e quantitative circa la progressione nel 2006 nella realizzazione del Mercato unico europeo e nella partecipazione ad esso dell'Italia. Mancano altresì Mancano altresì adeguate valutazioni qualitative e quantitative circa l'evoluzione verificatasi nel 2006 della competitività dell'Unione Europea (e in essa dell'Italia) nei confronti di Stati Uniti, Giappone, Cina, Russia, India. Quest'ultima mancanza è particolarmente grave, data l'estrema rilevanza del processo di globalizzazione delle economie in atto in tutto il mondo. Auspichiamo che nella prossima relazione annuale si ponga rimedio a queste carenze. Ed ora due parole di commento a quella che è forse la grande novità della politica dell'Unione Europea nel 2006, la «nuova politica energetica», annunciata con enfasi in varie occasioni e succintamente presentata alle pagine pagine 227-233 della Relazione. Tale politica si basa sostanzialmente sulla convinzione che la responsabilità del riscaldamento globale in atto sia dovuta principalmente alla emissione nell'atmosfera di anidride carbonica dovuta ai processi di combustione dei combustibili fossili, petrolio, carbone e gas naturale, effettuata dall'uomo negli ultimi 250 anni. È una convinzione condivisa dalla maggioranza degli scienziati del clima, ma non da tutti. In effetti lo stesso IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dell'ONU segnala nei suoi rapporti che l'uomo sta perturbando il clima non solo con l'emissione di anidride carbonica nei processi di combustione, ma anche con l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, la deforestazione, l'utilizzazione a fini irrigui di acque di fiumi e laghi, la creazione di enormi aree urbane, l'immissione nell'atmosfera di varie specie di aerosol, Ad esempio, la produzione del potente gas serra metano dovuta all'uomo, è valutata dall'IPCC aver avuto nel 2005 un effetto di riscaldamento sul clima pari a quasi un terzo dell'effetto dell'anidride carbonica da combustione. Ma la Commissione europea e l'Unione Europea non hanno dubbi: il riscaldamento globale in atto è tutto colpa della combustione dei combustibili fossili (che assicura l'80 per cento del fabbisogno energetico mondiale); tale combustione va quindi drasticamente e rapidamente ridotta. Al riguardo sono stati configurati a Bruxelles tre specifici obiettivi: primo, limitare il surriscaldamento della temperatura dell'atmosfera a non più di 2 gradi centigradi (rispetto alla temperatura media dell'era preindustriale); secondo, ridurre entro il 2020 l'emissione di anidride carbonica del 20 per cento rispetto alle emissioni del 1990 (obiettivo vincolante); terzo, incrementare le fonti rinnovabili fino a raggiungere entro il 2020 il 20 per cento del *mix* energetico complessivo (obiettivo per ora non vincolante). Ed ora alcune osservazioni. Circa il primo obiettivo, va innanzitutto sottolineato che nella storia del nostro pianeta la temperatura dell'atmosfera è sempre variata di qualche grado e non certo a causa dell'uomo. Senza scomodare le ricorrenti glaciazioni e considerando solo l'ultimo millennio, abbiamo avuto negli anni dal 1000 al 1300 un periodo più caldo dell'attuale, durante cui fu possibile la coltivazione della vite in Gran Bretagna e la colonizzazione da parte dei Vichinghi dell'attualmente ghiacciata Groenlandia Terra Verde), e negli anni dal 1550 al 1800 un periodo assai più freddo dell'attuale (definito Piccola glaciazione), caratterizzato, ad esempio, da sistematiche gelate del Tamigi. L'Unione Europea trascura questa variabilità naturale della temperatura dell'atmosfera e attribuisce alla combustione dei combustibili fossili tutto l'incremento di tale temperatura finora avuto a partire dall'inizio dell'industrializzazione (circa 1,1 gradi centigradi). È poi assai singolare che l'Unione Europea assuma un obiettivo come quello della limitazione a non più di 2 gradi centigradi del surriscaldamento della temperatura dell'atmosfera quando non si sa ancora in che modo questa temperatura dipenda dalle misure effettivamente assumibili. Perciò non si vede quali potrebbero essere i "provvedimenti" da adottare per garantire questa limitazione. I più moderni codici di calcolo riguardanti il clima della Terra non sono in grado di prevedere con sufficiente esattezza nemmeno la temperatura media dell'atmosfera che si determinerebbe se per un colpo di bacchetta magica da questo momento in poi cessasse l'emissione nell'atmosfera di anidride carbonica da combustione. Va poi sottolineato che questo obiettivo dipende (se e in quanto dipende) dal comportamento non solo dell'Unione Europea, ma di tutto il mondo. Qui l'Unione Europea esplicita una propria ambizione di *leadership* mondiale nella difesa dell'ambiente che pare veramente fuori posto. Quanto al secondo obiettivo, va segnalato che attualmente l'Italia emette una quantità di gas serra pari al 13 per cento in più di quella emessa nel 1990. Di qui al 2020, in 13 anni, l'Italia dovrebbe quindi diminuire le sue emissioni di anidride carbonica da combustione del 33 per cento! Ove si tengano presenti le notevoli inerzie dei sistemi energetici coinvolti e le oggettive limitazioni dei contributi che potranno derivare dalle politiche di risparmio energetico e di efficientizzazione

Simili considerazioni vanno fatte a riguardo del terzo obiettivo, che per fortuna non è considerato ancora vincolante. Attualmente le fonti rinnovabili rappresentano il 7 per cento circa del *mix* energetico totale. Pur con tutta la confidenza possibile sul futuro sviluppo dell'energia eolica, dati i costi ancora elevati del solare termodinamico e del solare fotovoltaico, anche questo obiettivo appare assolutamente non conseguibile. Anche solo questi brevi commenti, signor Presidente, evidenziano quale linea pericolosa abbia assunto l'Unione Europea nel settore energetico: una linea ispirata da discutibili convinzioni ambientalistiche, poco rispettosa delle diversità nazionali, sostanzialmente dirigistica, poco attenta alle conseguenze che l'aumento del costo dell'energia (da essa determinato) produrrà in termini di perdita di competitività dell'Europa nel processo di globalizzazione. Non ultime tra queste conseguenze una sensibile perdita netta di posti di lavoro e una non trascurabile diminuzione del livello di vita. Auspichiamo che il Governo intervenga a Bruxelles per indurre ragionevolezza e mitigare

Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, come ogni anno, e quest'anno quantomeno con ampio anticipo rispetto al solito, viene posta all'approvazione delle Aule parlamentari la legge comunitaria: l'atto con cui vengono recepite, nell'ordinamento legislativo del nostro Paese, le direttive comunitarie e con cui il Governo opera per sanare le procedure di infrazione aperte dall'Unione Europea nei nostri confronti. A giudicare dalla convocazione dell'Aula e dalla conseguente presenza che si registra, non si può non trarne un giudizio di scarsa attenzione e considerazione nei confronti di un provvedimento che costituisce invece uno degli atti più complessi e delicati che ogni anno il Parlamento si trova a varare e che, per impatto nell'ordinamento vigente, è probabilmente secondo solo al collegato disposto alla legge finanziaria. Molte infatti sono le materie oggetto di recepimento delle direttive comunitarie emanate che vengono interessate da questo provvedimento e che in diversi campi vanno a modificare e interessare la vita dei cittadini. Proprio al riguardo viene naturale una prima inevitabile riflessione: un provvedimento che spazia - com'è stato detto anche dal collega Stiffoni - dalla normativa sulla commercializzazione delle uova alla normativa di finanziamento sulle fonti rinnovabili, o dalla normativa per l'importazione del legname alla normativa sulla navigazione, o, ancora, dal recepimento dell'ordinamento giudiziario comunitario, in termini di cooperazione giudiziaria penale, agli svariati provvedimenti sulle politiche comuni nell'ambito dell'Unione Europea, quali il diritto societario e quello finanziario o fiscale, pone in sé la domanda, peraltro di non facile soluzione, di quale sia il contenitore, la forma e l'ambito più adeguato di applicazione e di recepimento delle direttive comunitarie. Il rischio più facile in cui si incorre, come a mio avviso in questo caso, è quello di una sorta di provvedimento *omnibus* che contiene in sé di tutto e di più, ma in cui scarsa è la consapevolezza da parte del legislatore circa l'impatto che il provvedimento determina nella realtà quotidiana e, conseguentemente, anche la percezione dell'importanza del provvedimento per il cittadino è probabilmente prossima allo zero. Questo perché carente è l'efficacia comunicativa che viene riservata a questi provvedimenti e ancor meno rimangono chiari alla pubblica opinione non solo i benefici, ma sovente anche la *ratio* che guida e presiede questi. Conseguenza di tutto ciò è, ormai da anni, la diffusa percezione in ambito di legislazione comunitaria, di una distanza che si fa sempre più ampia, anziché ridursi, tra i cittadini europei e le loro istituzioni. Tutto ciò nonostante la legislazione di settore abbia fatto notevoli passi in avanti verso un sistema di più efficace integrazione del nostro ordinamento legislativo con quello comunitario. Dalla legge La Pergola in poi, infatti, passando per la legge La Loggia di recepimento del nuovo ordinamento istituzionale avvenuta con la modifica al Titolo V della Costituzione e, in ultimo, alla legge Buttiglione con le novità introdotte sul piano procedurale e provvedimentale, si può dire che il legislatore nel nostro Paese si è dotato di un quadro organico di norme in grado di recepire adeguatamente le direttive comunitarie emanate nel nostro complesso sistema ordinamentale e di smaltirne progressivamente il pregresso inerente le procedure d'infrazione che risultano ancora aperte. Un atto, quindi, la legge comunitaria, che si trova costretto tra la necessità di fare presto, per assolvere nei tempi richiesti alle direttive emanate o per sanare le procedure d'infrazione aperte, e la necessità di fare bene per inquadrarle in maniera armonica nel nostro articolato ordinamento istituzionale. In questo senso meriterebbe una più seria riflessione l'opportunità di prevedere in futuro una vera e propria sessione parlamentare sulla comunitaria, per un esame adeguato alle materie oggetto di revisione normativa e per una discussione di vero orientamento del Parlamento nei confronti del Governo sulle posizioni da assumere per l'Italia nella fase ascendente dei provvedimenti, come la Relazione allegata alla legge prevede e richiede. Tra l'altro è degno di sottolineatura il fatto che la legge comunitaria 2007 introduce anche alcune modifiche alla recente legge Buttiglione riguardanti significative novità in termini di recepimento delle direttive, proprio all'insegna di una loro maggiore armonizzazione ordinamentale ed efficacia applicativa. Tali novità possono essere riassunte nell'autorizzazione al Governo a recepire le disposizioni attuative adottate dalla Commissione tramite regolamento, nell'obbligo per il Governo di comunicare al Parlamento gli atti comunitari posti a base dei propri atti normativi e nel fatto che il termine di delega legislativa, come ricordava il presidente Manzella, debba coincidere, di norma, con la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive e che sia, invece, di 90 giorni nel caso in cui lo stesso termine sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Significativo è stato anche il lavoro svolto dalla 14a Commissione nell'apporto all'esame del provvedimento, avendone modificato sensibilmente l'articolato normativo. La legge comunitaria constava infatti di 22 articoli quando fu presentata dal Governo al Senato e consta adesso, nell'atto predisposto dalla 14a Commissione, di 34 articoli, ciò a seguito di abrogazioni di parti significative del testo originario, come ha segnalato il relatore, ma anche a seguito di ampie e significative aggiunte intervenute. Le stesse 16 direttive in esame sono uscite, dall'esame della 14a Commissione, diversamente riarticolate nei due allegati A e B con una maggiore prevalenza a vantaggio dell'articolato B, con la previsione quindi da parte del Governo, negli atti di recepimento, dell'emanazione di decreti legislativi per i quali sia necessario il successivo parere parlamentare. Un aspetto su cui si è particolarmente determinata l'attenzione dell'azione di Governo è quello della riduzione dello *stock* di procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese da parte dell'Unione Europea. Al 31 dicembre 2006 risultavano ancora aperte 227 procedure di infrazione, di cui 188 per violazione del diritto comunitario e 39 per mancata trasposizione delle direttive stesse; erano però 275 le procedure di infrazione aperte ereditate da questo Governo e l'obiettivo di scendere sotto la soglia delle 200 procedure di infrazione entro la fine dell'estate, come ha recentemente dichiarato il Ministro, sembra, anche alla luce del provvedimento che stiamo esaminando, un obiettivo possibile e indubbiamente significativo di un direzione di marcia assunta da questo Governo di cui occorre obiettivamente dare merito. Da segnalare, tra l'altro, il dato, non privo d'importanza, che la gran parte delle procedure di infrazione aperte riguarda prevalentemente le materie di natura ambientale, a dimostrazione di come i temi complessi facciano più fatica ad uniformarsi nell'ambito della nostra legislazione specie laddove la nostra Costituzione prevede ormai una competenza concorrente tra Stato e Regioni. Una riflessione a sé merita senz'altro la Relazione della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, specie rispetto ai recenti sviluppi determinati dal Consiglio europeo di Bruxelles inerenti la spinosa questione del Trattato costituzionale. La Relazione costituisce parte integrante della legge comunitaria e fissa la cornice in cui si svolge l'azione di governo del nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea: in pratica, nel consuntivo - lo diceva molto bene il Presidente è implicito l'atto d'indirizzo che il Parlamento consegna al Governo, in specie per la fase ascendente dei provvedimenti. La Relazione si articola in cinque parti. La prima parte tratta delle questioni di stringente attualità, dal processo di integrazione europea alle questioni istituzionali, dalle questioni inerenti le relazioni esterne all'Unione Europea alla cooperazione interna nei settori della giustizia e della politica di sicurezza; particolare risalto viene dato alle questioni connesse alle politiche economiche, con riferimento al rilancio della crescita e della competitività.

parte della Relazione costituisce un'attenta disamina dello stato dell'arte circa le procedure di infrazione aperte, con l'elenco e i motivi, per la prima volta, delle impugnazioni e l'efficace strategia che questo Governo si è dato per ridurre lo *stock* di infrazioni all'insegna della costruzione di una posizione unitaria, migliorando le procedure di coordinamento istituzionale e in grado quindi di rafforzare la capacità negoziale del nostro Paese con l'Unione Europea. La terza parte illustra le linee evolutive delle tematiche relative al mercato interno dell'Unione Europea, che tradizionalmente si concentrano nell'integrazione e nell'apertura dei mercati. Un mercato interno che fornisce una scelta ampia di beni e servizi di qualità e con un'adeguata garanzia di protezione per il consumatore. Il completamento del mercato interno dovrà puntare al potenziamento e all'effettiva integrazione delle infrastrutture, a partire dai grandi corridoi transeuropei, unitamente ad una comune politica energetica e per l'ambiente, prospettiva questa cui il nostro Paese guarda con particolare interesse. La quarta parte illustra le linee evolutive relative alle politiche comuni. La quinta, infine, analizza l'andamento delle politiche economiche e dei flussi finanziari provenienti dall'Unione Europea all'Italia in relazione alle politiche di coesione sociale e della loro utilizzazione. Tornando in conclusione al recente Consiglio europeo di Bruxelles sul Trattato costituzionale, molto è stato detto e scritto circa il giudizio sull'approdo a cui è giunto e difficile è supporre possa essere detta una parola definitiva in proposito. Certo è che probabilmente si tratta di uno di quei casi in cui la soddisfazione o l'insoddisfazione non può che essere espressa solo a metà e che quindi nel giudizio pesano inevitabilmente molto di più le aspettative di ognuno che la reale valutazione del risultato conseguito. Soddisfazione deve essere necessariamente espressa per la rimozione di uno stallo in cui era precipitata l'Unione Europea dopo i *referendum* francese e olandese e a cui si erano assommate le resistenze del Regno Unito e le pervicaci ostinazioni dei cosiddetti Paesi euroscettici, primi tra tutti Polonia e Repubblica Ceca. Era inevitabile che la rimozione di questi ostacoli, peraltro non banali, pesasse comunque sull'esito finale e così indubbiamente è stato, non tanto per gli aspetti nominalistici o simbolici venuti meno rispetto a quanto era contenuto nel Trattato costituzionale, a partire dalla stessa definizione di Trattato costituzionale o alla bandiera e all'inno, quanto piuttosto per gli aspetti di sostanza che comunque nell'immediato risultano almeno in parte compromessi, a partire dalla modalità di voto a maggioranza, che di fatto viene rimandato al 2017 subendo così il ricatto assurdo della Polonia; o all'Alto funzionario (si spera non solo per statura fisica) in vece del Ministro degli esteri unico per l'Unione Europea, nell'interesse evidente della politica estera britannica; e, per finire, con la soppressione dagli obiettivi dell'Unione del riferimento al libero mercato e alla concorrenza non falsata, tanto cara al nuovo presidente francese Sarkozy, che ne aveva fatto un punto irrinunciabile nella sua campagna elettorale. Del resto (lo diceva anche il presidente Manzella), le politiche di libero mercato e di apertura alla concorrenza scontavano già da tempo ritrosie e ripiegamenti significativi, sicuramente da parte della Francia, ma che anche nel resto dell'Unione avevano suscitato più paure che un approccio di sfida all'insegna della concretezza e del pragmatismo nell'interesse generale del singolo cittadino. Indubbiamente il fattore tempo registra sfasature più lunghe di quanto gli europeisti convinti speravano e credevano; e, d'altra parte, il tempo in un processo di integrazione di così vasta portata e di così grandi ambizioni non può certo essere ridotto ad una variabile secondaria per la stessa Unione Europea, che ha fatto degli appuntamenti con le scadenze un proprio tratto distintivo e peculiare rispetto alla gran parte degli Stati membri, ma evidentemente non ancora un fattore unificante. Al di là della sostanza, che comunque resta presente nell'accordo raggiunto, il rischio vero che si apre per il futuro è quello di fare involvere il processo di integrazione europeo verso una semplice rete intergovernativa regolata dal vecchio gioco delle alleanze con i relativi rapporti di forza, anziché farlo evolvere verso un grande Stato federato, vero obiettivo sotteso al Trattato costituzionale. Certo è che l'Europa rimane uno straordinario progetto politico, l'unico che dal dopoguerra ad oggi ha garantito la diffusione di pace e benessere per una quantità crescente di cittadini che non si definiscono ancora europei, ma che sono ormai accomunati da una molteplicità di fattori caratterizzanti la vita quotidiana di centinaia di milioni di persone.

L'accordo raggiunto, per quanto parziale, è comunque un successo in quanto sblocca un'*impasse* che stava determinando una stasi pericolosissima. Del resto, verrebbe da dire che non c'è vero successo senza travaglio e non si costruisce il futuro rimuovendo il passato, ma soltanto facendo con esso i debiti conti, i conti mai facili della storia, come appunto in questo caso è stato fin troppo eloquente. Se quindi l'Europa ha vinto la propria sfida con la storia decretando, ancora una volta, che non c'è alternativa alla composizione degli interessi, è però a poco a poco divenuto sempre più chiaro che, come ha scritto Arrigo Levi, c'è anche un'altra sfida della storia ed è quella della storia futura, e questa è ancora tutta da vincere. In questo senso, possiamo dire che gli obiettivi di fondo dell'integrazione europea rimangono solidi rispetto a quelli di cinquant'anni fa: la pace, la prosperità e il miglioramento della qualità della vita di tutti gli europei rimangono un punto fermo come la stella polare. Appare però evidente, allo stesso tempo, che quegli obiettivi impongono la necessità di passare da un'Europa che guarda dentro di sé ad un'Europa che guarda sempre più fuori di sé, capace di intervenire con autorevolezza sulla scena mondiale maturando consapevolmente l'ambizione di governare i processi di globalizzazione, piuttosto che farsi governare da questi.

Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge comunitaria è l'occasione che annualmente ci si presenta per una riflessione dedicata al ruolo e allo stato della partecipazione dell'Italia al processo di costruzione europea. Due i grandi assi di interesse: il primo, il processo di integrazione europea in termini generali; il secondo, come l'Italia partecipa a questo progresso, come si organizza al proprio interno, cosa fa per sviluppare la conoscenza e la coscienza dell'Europa negli apparati e nei cittadini, come adegua il proprio ordinamento alle decisioni europee, quanto è stato fatto e quanto resta ancora da fare. Sul primo punto, ho già avuto l'onore di esprimermi in quest'Aula poche settimane or sono, quando abbiamo celebrato il 50° anniversario dei Trattati di Roma. Basta ricordare le difficoltà che ha incontrato e ancora incontra il percorso costituzionale dell'Europa, pur a fronte di un'esigenza incontestabile di un rapido, quanto profondo, consolidamento dell'Unione: proprio nel momento in cui l'Europa è cresciuta ha bisogno di visibilità e credibilità sulla scena mondiale. L'accordo al ribasso raggiunto faticosamente dai 27 rappresenta comunque una onorevole uscita dall'*empasse*, tanto da essere considerata da qualcuno come un grande progresso. Credo che occorra essere ottimisti. C'è bisogno degli europei perché l'Europa avanzi, c'è bisogno che i cittadini partecipino all'Europa e la sentano come un loro spazio istituzionale, perché l'Europa si rafforzi e non sia un mero affare di politica economica. Avvicinare all'Europa i cittadini, permettere ai cittadini e alle Regioni di agire in Europa e per l'Europa affinché l'Europa mantenga e rafforzi la sua vitalità. Vengo al secondo punto, relativo a come l'Italia partecipa al processo di integrazione. Già dalla relazione annuale presentata dalla ministro Bonino si evincono elementi di grande interesse, che riferiscono gli sforzi fatti per una politica dell'Europa che sia realmente partecipata da tutti gli italiani, più vicina ai cittadini e ai loro bisogni; una politica che sia coerente con gli impegni assunti e aperta ad un rafforzamento dell'Unione sulla scena internazionale. Ed anche il disegno di legge comunitaria per il 2007 testimonia di apprezzabili risultati e significative innovazioni: la progressiva riduzione dei tempi per il recepimento delle direttive e una maggiore attenzione per l'adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede comunitaria sono certamente segnali di rilievo, nel senso dell'efficienza e della serietà della posizione italiana. Così come è di assoluta importanza quanto previsto all'articolo 5, che delega al Governo l'emanazione di testi unici e, novità, di codici di settore al fine di coordinare nelle singole materie il complesso normativo di riferimento. Maggiore chiarezza nella normativa permetterà sicuramente un migliore e più immediato rispetto delle disposizioni. Da sottolineare infine la parte del disegno di legge, che interviene in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria, concorrendo a rinsaldare il cosiddetto terzo pilastro dell'Unione Europea. Condivisibile, dunque, l'impianto della legge comunitaria del 2007, nel suo contenuto complessivo e nella sua architettura. Permettetemi ora quale rappresentante di una Regione autonoma e del Gruppo Per le Autonomie qualche riflessione per quanto concerne il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle fasi ascendente e discendente del diritto europeo. Certo, attraverso le norme, questa partecipazione pare garantita. E in questo ambito molto è stato fatto. O meglio, è stato soprattutto scritto e detto, perché da fare, nel concreto, rimangono ancora alcuni passi decisivi. Mi riferisco alla partecipazione dei rappresentanti regionali al Consiglio dei ministri dell'Unione, nell'ambito della delegazione italiana, che attende di essere definita e pienamente attuata. Mi riferisco ad una fase ascendente, che veda l'effettiva e costante possibilità per le realtà territoriali, attraverso un loro continuo e serio coinvolgimento di seguire la nascita e lo sviluppo delle decisioni in sede europea e di potervi incidere tangibilmente, non solo di osservare e di esserne i passivi destinatari. Le articolazioni della Repubblica devono essere veri attori del processo comunitario; portatori degli interessi, dei bisogni, delle aspirazioni e delle esperienze delle rispettive comunità. Solo così è possibile diffondere la coscienza dell'Europa; solo così è possibile ridurre il *deficit* democratico che ancora segna il processo di integrazione. Penso, in ultimo, ad una fase discendente che deve essere l'occasione per le Regioni e le Province autonome di esplicare le loro competenze e la loro autonomia, in un quadro di riferimento chiaro, che non alimenti i contenziosi, siano essi innanzi all'Europa o in sede costituzionale. Comprensibile e opportuna la clausola di cedevolezza prevista dalla legge n. 11 del 2005 e dalla legge comunitaria; necessaria, perché l'Italia risponda con coerenza e serietà agli adempimenti comunitari. Ma non certamente uno strumento di cui abusare, perché comunque impattante ed invasiva. Meglio sarebbero una maggiore sensibilizzazione, più sollecitazioni preventive, una previsione efficace dei princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome debbono esercitare la propria competenza normativa. Sono punti e criticità dei quali la relazione del ministro Bonino ben rende conto e sui quali traspare l'impressione di un'accresciuta attenzione del Governo per una loro soluzione, e questo ci fa ben sperare. Credo che, in estrema sintesi, la ricetta stia nel raggiungere un elevato livello di concertazione politica e di leale collaborazione tra tutti i livelli di Governo. Ogni soluzione passa attraverso il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di autonomia. Un rispetto che, in processi complessi quali sono quelli europei, non può non incardinarsi su di un'effettiva quanto proficua partecipazione, che dal cittadino arrivi all'Europa, attraverso le diverse articolazioni della nostra società e gli enti territoriali. Questo perché l'Europa sia vissuta e sia sentita perché l'Europa cresca e si consolidi veramente con l'apporto di tutti e non rimanga una questione degli Stati o dei gruppi di interessi economici; perché l'Europa si sviluppi grazie alle proprie differenze, e non sia portatrice di appiattimento e di uniformizzazione; perché sia attenta alla qualità e alla condivisione delle sue decisioni, più che alla quantità e all'arricchimento dei mercanti. Ho apprezzato il fatto che l'articolo 7 del disegno di legge sia stato soppresso; una misura questa che avrebbe avuto l'obiettivo di favorire lo sviluppo del mercato a scapito dei produttori di qualità i cui interessi possono assolutamente coincidere con gli interessi dei consumatori: se questa è la strada che vogliamo seguire, non penso che siamo orientati verso un'Europa più coesa, ma solo verso un'Europa più uguale al suo interno, adagiata sul compromesso al livello più basso. E questo mi desta qualche perplessità, perché non corrisponde alla mia idea di Europa, fondata sulle differenze. Non corrisponde all'idea dei Padri dell'Europa, che volevano unire senza cancellare le diversità che anzi vedevano nell'equilibrio delle diversità, nella loro armonizzazione, la ricchezza dell'Europa. Non è questa un'Europa di buon auspicio per la salvaguardia delle sue specificità regionali e territoriali, attenta ai suoi cittadini, a quei cittadini e a quelle realtà territoriali che, invece, soli possono garantire il pieno successo del progetto europeo. E ciò un po' mi preoccupa, perché non mi sembra in linea con il riconoscimento delle specificità, quelle, per esempio, dei territori montani e dei prodotti di qualità, che invece considero come esigenze irrinunciabili. Mi sembra uniformizzazione, più che armonizzazione. Attenzione, però, perché uniformare crea resistenze e conflitti, non fa bene all'Europa, mentre armonizzare, condividere il percorso e il risultato, ascoltare le diverse esigenze e fare tesoro delle diverse esperienze è garanzia di successo, di vera coesione. Ma per fare ciò, dobbiamo poter partecipare; e per partecipare dobbiamo esserci.

Il diritto di partecipare all'Europa per una comunità come quella valdostana, alla quale è riconosciuta un'autonomia speciale, che è minoranza costituzionalmente tutelata, che è francofona e germanofona, che incardina i bisogni e le aspirazioni di una realtà di montagna e frontaliera, è sacrosanto. Vogliamo uguaglianza, vogliamo vedere infine riconosciuto questo diritto democratico ad essere presenti in Europa. Ogni Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma deve avere almeno un proprio rappresentante al Parlamento europeo, per concorrere alle decisioni, apportando il proprio contributo di realtà peculiare, per comprendere le esigenze dell'Europa e per presentare le proprie esigenze all'Europa. Urge un deciso e forte intervento del Governo e del Parlamento in tal senso, perché nessuno si senta escluso dall'Europa. Perché l'Europa non sia un rischio, ma sia un'opportunità per tutti. Signor Presidente, la presentazione di un ordine del giorno mi consente di svolgere alcune considerazioni, soprattutto sulla comunitaria e anche sulla relazione annuale che viene presentata, relativa alla partecipazione dell'Italia al processo di costruzione europeo. Ora, positivamente le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, che ha in qualche modo ripreso la strada di un cammino che sembrava interrotto; la determinazione della cancelliera

Devo lamentare, per esempio, i ritardi nell'esame del provvedimento che ho predisposto in occasione della celebrazione del progetto Antartide, come occasione per il rilancio della ricerca in quel continente.

L'Italia è in prima linea in questo settore, dispone di *know-how* adeguato e svolge un ruolo fortissimo nell'innovazione, soprattutto negli uomini, nelle risorse e nelle tecnologie.

per così dire, un'attenzione particolare. Ho presentato pertanto l'ordine del giorno G100, richiamando l'attenzione del Ministro delle politiche comunitarie nella prospettiva della Conferenza intergovernativa ESA che si terrà nel novembre 2008. si tratterà di un'occasione importante, in vista proprio delle definizioni dei compiti nell'esplorazione spaziale connessa con i nuovi impegni di spesa a carico dei vari Stati membri,

soprattutto a rappresentare il quadro finanziario rispetto al consolidamento del programma europeo di esplorazione e a definire nell'informazione sul piano strategico di settore, da concludere entro questo anno, non trascurando di accennare ai documenti programmati che sono previsti. chiarire soprattutto l'opinione del Paese rispetto alle seguenti parti integranti del piano strategico: il completamento della missione EXOMARS, le tecnologiche abilitanti per l'esplorazione Luna e Marte, da realizzare attraverso dimostratori strategici e tecnologici, le basi cooperative del veicolo trasporto umano CSTS e l'utilizzo della stazione spaziale per missioni di esplorazione. Tutto ciò lo abbiamo visto e lo vediamo progressivamente realizzato, però è necessario che la manifestazione di volontà del Governo, in ordine alle decisioni della Conferenza intergovernativa del 2008, rispetto al ruolo delle aziende italiane impegnate nel settore, alla conferma delle *leadership* già conseguite e alla presenza nei programmi per tecnologie abilitanti, abbia una definizione certa. Presidente, signor Ministro, ho presentato anche una proposta di legge in questo senso, per far sì che ci sia una definizione di coordinamento, perché la politica spaziale troppo spesso viene frammentata attraverso una serie di competenze. Occorre che la voce del Governo italiano sia una e, soprattutto, che si individui il tavolo rispetto al quale le varie questioni e i vari interessi possano in qualche modo convergere. Abbiamo la necessità di confermare tale volontà, di confermare l'impegno dei Ministri italiani per assicurare, attraverso apposite iniziative, la partecipazione creativa delle piccole e medie imprese ad alta definizione tecnologica, sia aerospaziale sia di altra natura, perché ciò ha fortissime ricadute nell'ambito della struttura produttiva del nostro Paese. Aggiungo un'altra considerazione. Siamo molto preoccupati per quanto riguarda la vicenda "Galileo" e abbiamo visto i ritardi che si sono realizzati rispetto alla partecipazione italiana,

se si mettesse in moto una domanda pubblica molto forte, soprattutto da parte delle amministrazioni regionali e comunali per i riflessi che ha quel progetto rispetto a prospettive di sviluppo e anche alla qualità della vita dei cittadini. Riteniamo che debba essere compiuto ogni sforzo affinché quel progetto possa essere rivitalizzato, unendo anche le considerazioni che ho esposto sulla politica spaziale, perché siamo protagonisti in tal senso. le decisioni che gli altri Governi e gli altri Paesi stanno portando avanti rispetto alle politiche spaziali per comprendere le ricadute che si determineranno. Voglio ricordare in particolare l'impegno che stanno portando avanti Paesi emergenti come la Cina e l'India, mentre si registra un ritardo, ad esempio, per quanto riguarda la vecchia Unione Sovietica, e quindi la nuova Russia,

Naturalmente in campo mondiale c'è una spinta dei Paesi a riprendere con vigore questi programmi, proprio per le ricadute che determinano sull'economia. Per queste ragioni mi auguro che l'ordine del giorno da me presentato possa essere accolto da parte del Governo, del ministro Bonino, per dare un segnale chiaro rispetto a queste politiche e, soprattutto, rispetto agli impegni che devono essere portati avanti. Lo stesso appello rivolgo al presidente Manzella

questa legge comunitaria ci conferma l'impressione che siamo sempre, come Paese e come legislatori, impegnati in una perenne ed affannosa rincorsa di quanto Bruxelles ci propone e ci impone. evidente come la mole di provvedimenti che piovono dall'Unione Europea è addirittura superiore alla capacità di recepimento di questo povero Paese. Non si spiegherebbe altrimenti come ci ritroviamo tutti gli anni a discutere di leggi comunitarie che non solo toccano la più vasta gamma di argomenti, come è prevedibile che sia, ma che comprimono, soffocano e nascondono provvedimenti che, per l'impatto destinato ad avere sul nostro sistema normativo, meriterebbero spazi dedicati, attenzione altissima, tempi di discussione più ampi, un *iter* insomma che non può essere definito solo dalla necessità di far presto per non essere bacchettati dalla Commissione europea. Posti di fronte ad una legge comunitaria che pone banane e fiori sullo stesso piano delle sentenze penali, al di là del rischio di cadere nel ridicolo, come parlamentari siamo anche oggettivamente limitati nella nostra funzione di confronto e di critica alla proposta governativa: approfondire e, se necessario, ostacolare alcune parti del provvedimento rischia di creare ritardi e porre a rischio di infrazione anche il recepimento di normative proporzionalmente più semplici e assolutamente necessarie e condivise. La mia critica non è diretta allo strumento della legge comunitaria in sé e per sé, che può essere anzi strumento ottimo, come ho detto, per tutti quei provvedimenti legislativi a carattere in gran parte tecnico che non sollevano questioni di opportunità politica o questioni di principio. Ma molto sta al buonsenso e, aggiungerei, alla buona fede del Governo che presenta il disegno di legge, nel non creare calderoni improponibili che oltretutto creano comunque ritardi problematici. Sarò pessimista, ma ho il forte dubbio che anche quest'anno il Parlamento non riuscirà a trasformare in legge la comunitaria prima dell'autunno. È assurdo, se pensiamo che il disegno di legge dovrebbe essere pronto a fine gennaio e che contiene termini stretti legati alla scadenza dei provvedimenti da recepire. Dunque, nel tentativo dì far passare piccoli e grandi granellini in un'unica valanga si finisce con l'ingorgare tutto. La nostra posizione sul disegno di legge comunitaria sarà fortemente condizionata dal dal mancato ascolto da parte del Governo dei nostri richiami ad un maggior ordine legislativo, con lo stralcio dal provvedimento generale di quei temi che per delicatezza e complessità meritavano un *iter* dedicato, nelle Commissioni competenti e con maggiori tempi di analisi: mi riferisco, logicamente, alla parte inerente i problemi della giustizia. Certo è che discutere oggi di normativa sfornata da Bruxelles, all'indomani di un Vertice europeo che ha intravisto il completo stallo del progetto europeo, lascia un po' di amarezza. Persino i *big* europei che dopo l'accordo *in* *extremis* hanno parlato di «bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno» lo hanno detto con facce ben poco convincenti. Ed infatti i giornali di tutta Europa non hanno risparmiato espressioni come "fallimento" e "accordo al ribasso". L'Europa che non ha mai avuto una Costituzione dieci giorni fa ha rinunciato per sempre ad averla. Qualunque cosa si partorirà nel prossimo futuro non sarà che un altro trattato che spiega le regole del gioco, i criteri di voto, le maggioranze e i poteri di ricatto, ma nessun documento che fondi su basi diverse, politiche o identitarie, l'Europa nata dal mercato. Tutti i pronostici da noi sostenuti nel corso degli anni si sono purtroppo realizzati: l'Unione dei tecnocrati nulla ha compreso del sentimento dei cittadini, con il risultato che sono riemersi egoismi nazionali e, addirittura, velleità di chiusura e isolamento nazionale. II libero mercato, portato alle sue estreme conseguenze, ci ha esposti a una concorrenza selvaggia, deleteria per il nostro sistema produttivo, tanto che la grande Francia europeista ha posto un freno pesantissimo alla concorrenza, lasciando intendere che non esiterà a proteggere con tutti i mezzi i propri campioni industriali nazionali. È uno schiaffo al vice presidente della Convenzione Europea che elaborò la bozza di Trattato costituzionale, Giuliano Amato, e all'allora presidente della Commissione, Romano Prodi, che si erano battuti invece perché la libera concorrenza entrasse di peso nel Trattato, nonostante i tanti pareri contrari giunti durante il lavoro della Costituente. Dall'altro lato, abbiamo i Paesi di recente adesione che, confermando ancora una volta la tesi della Lega, non hanno certo chiesto l'ingresso nell'Unione per recitare la parte degli *yesmen* eternamente grati alla vecchia Europa per la bontà con cui li ha accolti tra le sue mani caritatevoli. Questi Paesi, con un passato tragico che ancora brucia, non sono guidati da fanatici, ma da grandi calcolatori. Nell'Unione pestare i piedi, rivendicare pretese al limite della provocazione, tirare la corda al massimo è una politica che paga: chi batte i pugni vince. Ce lo ha insegnato la Gran Bretagna, che con i suoi continui distinguo gode ancora di privilegi vecchi di venti anni, beneficia di autonomia decisionale e monetaria e, solo quando le fa comodo, fa proprie le normative europee. Londra, infatti, ha preteso e ottenuto nell'ultimo Vertice che la giurisprudenza inglese non debba soggiacere a quella europea: l'esatto contrario di quanto facciamo noi con questa comunitaria in tema di giustizia. La Polonia ci ha insegnato nello scorso *week end* che lo slancio idealista dei Padri fondatori è un malinconico ricordo, che va benissimo per essere citato negli anniversari, ma nella realtà deve lasciare spazio ai calcoli di opportunità e alle prove di forza. Questo lo scenario continentale. Ma il disastro generale non deve far passare sotto silenzio il nostro disastro casalingo, il ghetto dentro il quale sembra si stia gettando il nostro Paese. L'abbiamo detto mille volte: l'Italia, indipendentemente dal Governo che la regge, intontita dalla propaganda europeista che ha particolarmente attecchito nel nostro Paese, attua la strategia polacca al contrario: non batte mai i pugni sul tavolo, dice sempre di sì a tutto senza discutere; guai a non sembrare abbastanza idealisti e sognatori, guai che qualcuno ci dica che per colpa nostra l'integrazione non va avanti a spron battuto. Di ciò paghiamo le conseguenze su tutti i fronti: non nominiamo funzionari italiani nelle istituzioni, così che quando abbiamo bisogno di interlocutori dobbiamo imparare il lituano per farci ricevere; regaliamo il tocai, l'indotto e la tradizione vinicola appena qualche Paese ce lo chiede, e non certo per favore; versiamo a Bruxelles più soldi di quanto riceviamo come aiuti strutturali. Per una cosa del genere Londra, che sicuramente ha meno problemi di cassa di quanti ne abbiamo noi, riceve indietro i suoi soldi dai tempi della Thatcher. Ma da circa un anno l'Italia si fregia di avere un presidente di Commissione europea a capo del Governo. Che grande occasione! Giungendo direttamente dai vertici delle istituzioni comunitarie, probabilmente dal suo organo più potente dal punto di vista concreto, porta in dote grande prestigio e credibilità, nonché grande conoscenza dei meccanismi e degli strumenti, tale da rappresentare un ritorno in grande stile dell'Italia sulla scena europea (questo ci era stato contrabbandato). Non so quanti dei nostri concittadini sappiano che Prodi è stato tenuto alla porta di ogni riunione decisiva del Consiglio europeo. Oltre ad averlo visto nelle foto di rito, abbiamo letto dei ruoli giocati dalla Merkel, dai gemelli di Varsavia, da un Blair prossimo al ritiro e dal neoeletto Sarkozy. Pensate che durante la riunione finale e decisiva di questi *leader* il nostro Presidente del Consiglio era in un'altra stanza, ad ingannare il tempo con altre otto delegazioni considerate chiaramente minori. Da Paese fondatore e potenza mondiale a giocatore in panchina, in attesa delle scelte dei professionisti. Cosa ha rappresentato l'Italia in questo Vertice? Che contributo ha portato? Che parere è stato chiesto al Parlamento e ai cittadini riguardo al ruolo da sostenere? Che prospettive possiamo avere, in futuro, dentro l'Unione Europea? E perché il Presidente del Consiglio, senza battere ciglio, ha sottoscritto il pallido accordo uscito dal vertice europeo, dopo aver giurato e spergiurato che non avrebbe mai accettato compromessi al ribasso, facendo proprio il contrario di quello che aveva garantito al Presidente della Repubblica nell'incontro del 16 maggio scorso? Presidente, che figura da chiodi!

L'approvazione della legge comunitaria è nel nostro ordinamento un atto fondamentale per la costruzione di una concreta sintonia tra la legislazione nazionale e le diverse forme di decisione assunte in sede europea. Una sintonia che però ancora stenta ad affermarsi e a dispiegarsi completamente a causa di ritardi da attribuire alla lentezza ed alla viscosità dei processi, ma anche da attribuire ad un ritardo di natura più generale che riguarda tutti: alla modalità, cioè, di affrontare la questione europea più come pratica da sbrigare o magari da rinviare, secondo le diverse opinioni, piuttosto che come il vero nuovo orizzonte della politica. La debolezza del sistema di partecipazione nella fase ascendente, poi, determina spesso una conseguente resistenza nella fase discendente, quella di attuazione delle direttive e delle decisioni quadro, producendo così l'accumulo di un numero consistente di procedure d'infrazione. Il nostro Paese, che pure è considerato un Paese a forte vocazione europeista, naviga ancora agli ultimi posti di questa graduatoria, sia per il numero complessivo di infrazioni pendenti, sia per il numero di quelle aperte nel singolo anno. È quindi da accogliere come una positiva novità l'inversione di tendenza che finalmente si è determinata nel secondo semestre del 2006 con la diminuzione dalle 244 procedure d'infrazione di fine giugno alle 226 di fine anno. Un risultato importante, ma da ritenere non ancora sufficiente, che può essere certamente migliorato da procedure più snelle e razionali, dal rafforzamento di strumenti, quali la struttura di missione, che si sono dimostrati particolarmente efficaci, dal crescente coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali e della loro responsabilità diretta del rispetto della normativa, che troverà ulteriore giovamento anche dalle innovazioni che sono state introdotte in questa comunitaria relativamente ai tempi di attuazione delle deleghe, ma che soprattutto richiede un incremento significativo della partecipazione alla formazione delle scelte, tale da coinvolgere, in modo più efficace, tutti i luoghi della rappresentanza, a cominciare dai Parlamenti nazionali. Solamente la consapevolezza e la condivisione delle procedure e dei risultati di tali scelte possono rendere rapida ed efficace la loro successiva trasposizione nella legislazione nazionale e regionale e rendere quei princìpi patrimonio acquisito della pubblica amministrazione. La politica europea non è la politica estera, ma il nuovo ambito attraverso cui si realizza una parte sempre più consistente dell'intervento sulle condizioni sociali, ambientali ed economiche delle nostre popolazioni. Per questo la discussione sulla comunitaria e sulla Relazione non può essere separata né dal momento della verifica, né dalla discussione sulle prospettive dell'Unione e sul ruolo forte che essa può assumere di fronte alle nuove emergenze planetarie in quel grande catino in ebollizione in cui si alimentano reciprocamente guerre e terrorismo, dove la crisi ambientale e gli squilibri sociali mettono a rischio la centralità della persona, del suo lavoro e della sua piena inclusione sociale, un sistema di valori proprio del vecchio Continente che si è progressivamente definito nelle diverse epoche attraverso la cultura classica, il pensiero cristiano, l'umanesimo, le rivoluzioni borghesi, le istanze e le conquiste del movimento operaio. Pochi giorni fa si è concluso il Consiglio europeo di Bruxelles, dove si è discusso il destino del Trattato costituzionale, chiudendo la cosiddetta pausa di riflessione. Qui in Senato - dobbiamo dirlo - non siamo riusciti ad incardinare la discussione in tempi utili per affrontare quei temi prima di quell'appuntamento, per esercitare così il nostro ruolo di indirizzo che, pure nel rispetto delle competenze e nella attuale modalità delle relazioni comunitarie, costituisce l'espressione concreta e irrinunciabile del processo democratico. In particolare, in questo ramo del Parlamento siamo riusciti ad utilizzare ore ed ore per discutere - naturalmente in modo legittimo, signor Presidente - sull'ordine dei lavori, con varie e svariate polemiche, su tutte le questioni di maggiore o minore attualità, senza però riuscire ad affrontare questo tema e ad individuarne la centralità istituzionale e politica. A Bruxelles si sono registrati consistenti arretramenti. Sarebbe stato Sarebbe stato necessario superare l'ossimoro del Trattato costituzionale, abbandonando la forma del trattato e muovendo verso la costruzione condivisa di una autentica Carta costituzionale, che fosse capace di interpretare in positivo le istanze poste dalle bocciature referendarie e di mettere in moto il processo di costruzione democratica. Così non è stato. Anzi, si è abbandonata la strada della Costituzione e si è ripiegato definitivamente sulla forma del trattato; nemmeno di un nuovo trattato più o meno "mini", ma la semplice rivisitazione dei testi già in vigore. Per questo, per il poco coraggio nel raccogliere durante la "pausa di riflessione" le istanze insite nelle bocciature referendarie, alla fine hanno potuto brindare a Londra e a Varsavia, piuttosto che a Parigi e ad Amsterdam, per riprendere una espressione usata dal nostro Ministro degli esteri durante l'incontro con le Commissioni riunite affari esteri e politiche dell'Unione Europea. Una situazione che poteva andare anche peggio e, d'altronde, non c'è mai fine al peggio: è salvo il principio della personalità giuridica; è salvo, sebbene diluito nel tempo e nelle modalità di applicazione, il principio del voto a maggioranza; è salva, sebbene anch'essa indebolita, la figura del Ministro degli esteri attraverso una nuova e meno impegnativa definizione del suo ruolo come «alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza». Non andiamo avanti, dunque, anzi arretriamo; ma non tutti gli spazi sono chiusi per poter ripartire. C'è bisogno di un'Europa solidale dentro e fuori dai propri confini, di un'Europa che non si limiti all'integrazione dei mercati ed alla concorrenza, ma che sia capace di dare risposte alle vecchie e nuove emergenze rompendo il sistema della potenza militare come paradigma delle reazioni internazionali e dell'unilateralismo senza sostituirlo con un nuovo confronto tra blocchi contrapposti, ma attraverso la pratica e la proposta di una società organizzata intorno al primato del rispetto delle donne e degli uomini, del loro lavoro, della loro fatica, di modelli di relazione economici tra gli individui e tra gli Stati che non producano squilibri, ma che anzi possano attenuarli. Un'Europa che sappia scegliere e proporre altre strade per l'unico sviluppo possibile, quello compatibile con la difesa dell'ambiente e delle forme di vita che ospita. O l'Europa è all'altezza di questa sfida, o la sua necessità storica rischia di declinare irrimediabilmente. Per evitare questo esito la strada da percorrere è una sola, quella della democrazia: l'unica che possa costruire una comunità reale e che possa proporsi concreti obbiettivi di trasformazione. Mentre il senso comune è pervaso da nuove terribili incertezze ed esprime un grande bisogno di governo pubblico dei processi, i grandi mutamenti della globalizzazione ridislocano le scelte fondamentali per la vita delle popolazioni lontano dai luoghi della rappresentanza. Le tradizionali politiche nazionali perdono così di efficacia e di credibilità; i Governi, le istituzioni, la stessa politica appaiono lontani ed inutili. L'Europa può essere una risposta nuova e concreta, capace di essere alla altezza dei bisogni sociali emergenti, purché si fondi sulla ricostruzione di reali processi democratici. Ciò che fino ad oggi abbiamo sostenuto, a partire da un nuovo ruolo del Parlamento europeo entro cui si materializzi il percorso verso una vera fase costituente, non è stato archiviato dall'ultimo Consiglio, anzi crediamo si mostri oggi in tutta la sua ultimativa necessità.

ma come sarà possibile se le uniche notizie che hanno la forza di arrivare fino ad intrecciarsi con la materialità delle condizioni sociali sono l'aumento dei tassi di interesse decretato dalla BCE e la litania rigorista, spesso maliziosamente amplificata per appannare la diretta responsabilità di scelte economiche antipopolari e per tentare di impedire, attraverso questa via, che si dia corso a quell'impegno elettorale che abbiamo assunto con gli elettori ed unanimemente sottoscritto nel programma tra tutte le forze dell'attuale maggioranza? Mi riferisco alla rimozione di quello scalone che mortifica in un solo giorno le legittime attese di progetti di vita di tante donne e di tanti uomini giunti ormai alla soglia del trentacinquesimo anno di attività lavorativa. Abbiamo bisogno di una riforma della politica, di una riforma semplice: fare fare ciò che si dice e dire quello che si fa, null'altro. Questo già basterebbe a rilanciare il nostro ruolo e quello della stessa politica. Il Ministro degli esteri, per tornare alle nostre questioni, nella sua già ricordata relazione alle Commissioni riunite affari esteri e politiche ha richiamato la necessità di affrontare con realismo il dibattito ed il confronto sul futuro dell'Europa, pena la perdita di efficacia. È un richiamo giusto e condivisibile. Dobbiamo stare sul punto, ma mentre ci adoperiamo per influire sugli equilibri determinati dalle posizioni e dagli interessi dei singoli Governi, non possiamo non dichiarare la necessità di una lunga prospettiva, di una ricerca di senso, di significato. Quella prospettiva che ci può consentire di marciare a piccoli passi, magari su sentieri tortuosi, non sempre lineari, ma nella giusta direzione, quella di un'Europa dei popoli e della pace, una pace tra le persone, tra i popoli, tra l'uomo e l'ambiente; di un'Europa che sappia attingere alla più importante delle risorse, quella della democrazia e della partecipazione.

rispetto alle passate edizioni: da un lato, la previsione della coincidenza del termine della delega legislativa con la scadenza del termine di recepimento delle direttive contenute nel provvedimento; dall'altro, la previsione di disposizioni che danno attuazione, sempre mediante delega al Governo, a quattro decisioni quadro relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria, il cosiddetto pilastro dell'Unione Europea. A fronte di tali novità occorre registrare, però, la nota negativa relativa al fatto che l'impianto dell'intero disegno di legge, così come predisposto dal Governo, sia stato concepito facendo riferimento alla vetusta idea della legge comunitaria quale legge *omnibus*, ovvero atto legislativo che contiene una congerie di disposizioni volte a dare applicazioni a direttive comunitarie che toccano le più svariate e complesse materie. Una sorta di "treno" legislativo dove poter agganciare di tutto e di più, ossia qualunque genere di norma, dalle famose galline ovaiole, alle etichettature delle bevande, alla *golden share*, alle disposizioni contro l'Iran, all'importazione di legname e, infine, appunto, alla cooperazione di polizia e giudiziaria. Mi chiedo se questo sia il metodo più appropriato per affrontare materie delicatissime. Soprattutto, mi chiedo se questioni così complesse, che abbisognano di una ben più ponderata riflessione e di un più accurato approfondimento non debbano essere trattate, invece, in una sede diversa da quella dell'esame del disegno di legge comunitaria. Oppure, se non sia il caso che a tali problematiche, ancorché inserite nel disegno di legge comunitaria annuale, venga assegnato un tempo più congruo per essere proficuamente disaminate. Invece, netta è stata la sensazione, durante l'esame del provvedimento in Commissione, di un approccio superficiale e improvvisato da parte del Governo, che, più di una volta, attraverso emendamenti o subemendamenti fatti presentare dal relatore, ha introdotto nuove fattispecie al disegno di legge, in maniera caotica e, spesso, priva di coerenza. In tal modo, lo si è trasformato in un *corpus* eterogeneo ed affastellato di regolamentazioni, privo quindi di una visione unitaria che presupponga, invece, un approccio strategico circa la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, una visione non episodica circa il suo modo di essere nella trasposizione della normativa comunitaria nel nostro ordinamento. È legittimo parlare, in questo caso, di «riscrittura» del provvedimento, licenziato solo nel marzo scorso, attraverso l'innesto surrettizio di una miriade di nuove disposizioni riguardante ambiti del tutto imprevisti. Non credo che questo sia un modo lodevole di considerare il Parlamento, e, nel nostro caso, il Senato. Non credo neanche che questo sia il miglior modo di lavorare, perché si impedisce, di fatto, al *côté* parlamentare di esaminare con cognizione e con la dovuta cura materie primarie, che, soprattutto, toccano la vita di ciascun cittadino. A tutto ciò occorre aggiungere il *punctum* *dolens* riguardante la circostanza che il presente disegno di legge non risolve minimamente l'annoso problema delle infrazioni comunitarie. Come noto, l'Italia continua a rimanere il fanalino di coda per il numero di procedure avviate a suo carico per violazione del diritto comunitario o mancata trasposizione di direttive. Tale dato implica che lo Stato italiano ha un numero di infrazioni superiore a quello di tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea, compresi quelli di recente adesione all'Unione. Per l'esattezza, l'Italia, secondo l'ultima tabella aggiornata all'8 marzo scorso, figura al terzultimo posto per numero di direttive attuate, facendo meglio soltanto del Portogallo e della Romania. Secondo la relazione al disegno di legge, aggiornata al 31 dicembre 2006, inoltre, le procedure ufficialmente aperte sono complessivamente 227, tra le quali figurano 8 procedure ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. Queste Queste ultime discendono dalla mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, già passata in giudicato, e possono concludersi con l'irrogazione di una condanna che imponga il pagamento di una penalità o di un'ammenda forfetaria. A questo punto, non è possibile assolutamente sottovalutare il grave rischio che lo Stato italiano incorra in sanzioni pecuniarie, atteso che, in seguito alla sentenza del 12 luglio 2005 contro la Repubblica francese, nella causa C-304/02, la Corte di giustizia e la Commissione europea hanno adottato un nuovo orientamento, fondato sull'applicazione cumulativa dell'ammenda forfetaria e della penalità di mora (che possono arrivare anche fino a 700.000 euro al giorno), irrogabili anche qualora lo Stato adempia prima della seconda sentenza. In altri termini, esiste il rischio che lo Stato inadempiente venga condannato al pagamento di una somma forfetaria relativa al periodo intercorso tra la prima sentenza di condanna della Corte e il momento di effettivo adeguamento al diritto comunitario. A fronte di questa situazione fortemente preoccupante sarebbe stato almeno auspicabile riscontrare, nello stesso disegno di legge comunitaria, un maggior numero di disposizioni dirette a risolvere procedure di infrazione. Diversamente, si è preferito procedere percorrendo la strada «episodica» e occasionale degli interventi limitati e *ad hoc*, quando invece sarebbe stato necessario e indispensabile affrontare il problema delle infrazioni in maniera complessiva, cercando di risolverlo con meccanismi preventivi, permanenti e istituzionali, e, soprattutto, secondo un metodo che consideri l'insieme delle infrazioni imputate all'Italia come un *package deal*, ossia un pacchetto di inadempienze che occorre valutare principalmente per la potenziale ingente ricaduta finanziaria a danno dell'erario. Ci riserviamo quindi, signor Ministro, signor Presidente, in sede di approfondimento dei relativi emendamenti, di poter più dettagliatamente completare, laddove ci sarà consentito, il pacchetto di norme non valutato approfonditamente dal disegno di legge, sperando che con l'approvazione e anche con il parere favorevole del Governo alcuni emendamenti, soprattutto quelli sulla giustizia, potranno essere accolti con favore da parte non solo del Ministro, ma dell'intero Senato. Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signora Ministro, la legge comunitaria 2007, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee», contiene un insieme variegato di disposizioni e di fonti normative che hanno alle volte poco a che fare l'una con l'altra. Per altro, all'interno della cosiddetta legge comunitaria 2007 sono previste una serie di disposizioni in materia di giustizia e di lotta alla criminalità che presentano aspetti di novità e di sicuro rilievo. La Commissione giustizia del Senato ha già espresso formalmente un parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni all'insieme di queste disposizioni. Il mio intervento, perciò, si limita sinteticamente a commentare le norme in materia di giustizia e di lotta a varie forme di criminalità sia dal punto di vista giudiziario che da quello di polizia. Le norme in questione sono presenti negli articoli 18, 19, 20, 21 e 22. Le tematiche principali sono inserite nelle decisioni quadro comunitarie attinenti in particolare alla lotta contro la corruzione nel settore privato, provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, confisca di beni, strumenti e proventi di reato, applicazione del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. La prima decisione quadro da valutare è quella del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Voglio ricordare solo alcuni aspetti, facendo mie alcune considerazioni, per altro già emerse e approfondite in sede comunitaria. Vi si legge: «Insieme alla globalizzazione si è assistito negli ultimi anni ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. i casi di corruzione nel settore privato all'interno di uno Stato membro non sono più soltanto un problema nazionale, ma anche un problema transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un'azione comune a livello dell'Unione europea». A questo proposito va detto che gli Stati membri della Comunità hanno attribuito particolare importanza alla lotta contro la corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato, poiché ritenevano e ritengono che la corruzione in entrambi i settori abbia costituito e costituisca una minaccia innanzitutto allo Stato di diritto, anche generando distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali ed ostacoli per un corretto sviluppo economico. In tale contesto, non sono numerosi gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione europea del 1997 e del 1999 e quindi questo è uno dei punti che dovranno essere affrontati. Sempre a questo proposito, ricordo come in materia di lotta alla corruzione esista anche una convenzione ONU, sottoscritta dall'Italia nel dicembre 2003, e che ancora giace in attesa di essere ratificata dal Parlamento italiano, e in particolare in questo momento si trova agli atti della 3a Commissione del Senato. Il cuore della direttiva, per altro, che ci riguarda è rappresentato dall'articolo 2, che tratta di corruzione attiva e passiva nel settore privato: «Gli Stati membri - dice -adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali». E qui vengono indicate una serie di variegate fattispecie quali la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta, tramite un intermediario, di «un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere». Un'altra fattispecie, per altro molto ampia, è quella relativa alla lettera *b)*, dove si parla di «sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura,

per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere». Qui il riferimento alla violazione di un dovere è fatto in maniera chiara ed esplicita a quello che è l'interpretazione del diritto nazionale. La seconda decisione quadro, che si affianca a quella del 22 luglio 2003, reca la stessa data ed è relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di o di sequestro probatorio. Anch'essa è estremamente importante, soprattutto nella lotta alla criminalità. La premessa di questa decisione quadro è costituita da una deliberazione del Consiglio europeo deliberazione del Consiglio europeo del 1999 che aveva approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Lo scopo di questa decisione quadro è quello di stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, con una tutela specifica, prevista dalla decisione quadro, relativa ad un obbligo di tutela e di rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici fondamentali di cui all'articolo 6 del Trattato. Le figure di reato che sono rappresentate nella decisione quadro e che consentono un'applicazione del provvedimento di sequestro e di blocco vengono adottate ai fini probatori oppure per la successiva confisca dei beni. I reati per i quali sono previsti tali interventi sono quelli che hanno una punibilità nello Stato di emissione del provvedimento con una pena privativa della libertà di almeno tre anni. Non viene richiesto il controllo della doppia incriminabilità quando si tratta di reati particolarmente gravi: faccio sintetico riferimento ai reati che concernono il terrorismo, la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di bambini in pornografia, la corruzione, il traffico illecito di stupefacenti, di armi e di munizioni. Il dato fondamentale di questa decisione quadro è quello del riconoscimento di un'esecuzione immediata, perché viene esplicitato che le autorità giudiziarie riconoscono il provvedimento di blocco o di sequestro senza che siano necessarie altre formalità e viene adottata senza indugio la misura necessaria all'esecuzione immediata, alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, con alcuni limiti di tutela che sono quelli previsti dai principi fondamentali. fondamentali. Collegata alla decisione quadro del 2003 in materia di blocco dei beni è quella del 24 febbraio 2005, che concerne la confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Anche qui è evidentissima la finalità di contrasto alla criminalità, soprattutto a quella organizzata. Al riguardo alcune semplici considerazioni si impongono, perché la motivazione fondamentale, come è risaputo, della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sull'individuazione, il congelamento, il sequestro e la successiva confisca dei proventi di reato. Ciò è tuttavia ostacolato, tra l'altro, dalle differenti legislazioni in materia degli Stati membri. Un aspetto particolare parimenti noto è quello che deriva da una raccomandazione del 2000 in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata; una raccomandazione che riguarda il Consiglio europeo e che indica che occorrerebbe esaminare, proprio per favorire la lotta proprio per favorire la lotta alla criminalità organizzata, l'eventuale necessità di uno strumento che introduca la possibilità di mitigare (nell'ambito del diritto penale, civile o fiscale, a seconda dei casi) l'onere della prova per quanto riguarda l'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso con la criminalità organizzata. Non si tratta di una previsione o di una raccomandazione estemporanea, perché

della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che risale al dicembre 2000 e che prevede che le parti possano valutare valutare la possibilità di chiedere a chi abbia commesso un reato di documentare l'origine legittima dei presunti effetti o proventi confiscabili, sempre che tale richiesta sia compatibile con i principi del diritto nazionale e con la natura dell'autorità giudiziaria. L'articolo fondamentale di questa decisione quadro è quello che fa riferimento all'articolo 2 e prevede come ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di strumenti o proventi di reati punibili punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno, o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi. In particolare, va ricordato come ci sia una previsione esplicita anche per i reati di natura fiscale, in quanto per tale previsione, che va considerata positivamente, gli Stati membri possono ricorrere a procedure anche diverse dalle procedure penali per privare l'autore del reato dei proventi che ne derivano. L'ultima decisione quadro è anch'essa del febbraio 2005 e concerne l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Anche questa decisione quadro si rifà al Consiglio europeo dell'ottobre del 1999, che aveva sostanzialmente approvato il principio del reciproco riconoscimento, che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, tanto in materia civile, quanto in materia penale. Tale principio del reciproco riconoscimento dovrebbe applicarsi anche alle sanzioni pecuniarie comminate dalle autorità giudiziarie o amministrative al fine di facilitare l'esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state comminate. Importante a questo proposito è ricordare la definizione che viene data di sanzione pecuniaria, una definizione nuova, per una parte della quale mi permetto di sollecitare un ripensamento parziale da parte del relatore. Per sanzione pecuniaria si intende l'obbligo di pagare una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposto in una decisione dell'autorità giudiziaria; si riconosce l'obbligo di pagare una somma di danaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi; si intende l'obbligo di pagare una somma di danaro da versare a favore di un fondo pubblico di organizzazione e assistenza alle vittime, imposto nella stessa decisione dell'autorità giudiziaria. c'è una parte di questa definizione che deve, a mio avviso, essere ancora ampliata e che è quella relativa al concetto di risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, perché questa nuova definizione della decisione quadro, riportata poi pari pari, con rinvio, nell'articolo 34, del disegno di legge che dovremmo approvare, fa riferimento anche all'obbligo di pagare il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione dell'autorità giudiziaria, vengono però escluse

Per concludere, ricorderò soltanto che la Commissione giustizia ha valutato positivamente, in particolare, la previsione dell'obbligo del parere parlamentare su tutti gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega conferita al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta di materie notoriamente sensibili, anche molto sensibili, per le quali si ritiene importante che il Parlamento, in ragione proprio del carattere particolarmente delicato del tema, sia tempestivamente informato e possa puntualmente intervenire attivando i suoi ordinari poteri di controllo sull'operato del potere esecutivo. Signor Presidente, onorevole Ministro, credo che nell'analisi dettagliata della legge comunitaria avremo occasione, durante l'esame degli emendamenti, di fare alcuni approfondimenti. Ritengo che in questa discussione generale si debba affrontare il tema più ampio, il quadro, lo scenario nel quale ci stiamo muovendo: faccio riferimento alla risoluzione, presentata dai senatori Dini, Manzella, Zanone, che fa un po' la storia di una vicenda che si è conclusa - secondo noi - in maniera negativa a Bruxelles, alla fine della presidenza tedesca. Vi è stato un momento particolare nel dibattito avvenuto nel nostro Paese in merito alla Costituzione europea. E ricordo una risoluzione, presentata ed oggi correttamente abbandonata perché superata

ed anche indicato al Governo il modo nel quale era possibile, secondo noi, salvare il principio costituzionale, cercando di dare una diversa interpretazione all'architettura degli stessi trattati costituzionali, rendendoci conto che forse la Carta dei diritti poteva essere sganciata dal trattato stesso e come le leggi organiche di applicazione potevano aprirsi ad un confronto e ad un dibattito successivo. Purtroppo la vicenda non è andata come auspicavamo. Resta di fondo questo atto politico, che certamente rimane agli atti del Parlamento, un Parlamento così spesso diviso su molti argomenti, ma che sulla vicenda europea aveva ritrovato una sua unità di indirizzo; resta la delusione onestamente per quello che è avvenuto e per i risultati ai quali siano arrivati. È una delusione all'europea, nel senso che spesso si è delusi di come va l'Europa. Peraltro, giustamente si può anche dire che comunque un passo avanti, pur piccolo, lo abbiamo fatto e quindi in qualche modo l'Europa va avanti. Su questo modo di ragionare - che capisco, per cui apprezzo anche lo sforzo del presidente Manzella nella risoluzione, laddove cerca di individuare comunque gli elementi positivi che hanno

l'Europa. E non ci illudiamo nemmeno che l'avere ancora riconosciuto l'esistenza di un Alto rappresentante per gli affari esteri sia un successo. L'impegno era quello di arrivare ad avere una politica estera comune, addirittura un Ministro degli esteri comune! Siamo ancora molto lontani, e con tutto il rispetto per il signor Solana, che oggi è l'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'Europa, non credo che poter continuare nel modo in cui abbiamo operato fino ad oggi sia un passo avanti verso la costruzione di una politica europea. Allora, con grande serenità occorre prendere atto - all'europea - che questa è la realtà, che evidentemente esistono ancora molti Paesi che non hanno nessuna intenzione di rinunciare a quote di sovranità nazionale,

Noi non abbiamo mai parlato di allargamento verso l'Est dell'Europa: abbiamo sempre preferito parlare di riunificazione, proprio perché il *vulnus* che si era creato alla fine della seconda guerra mondiale, la cosiddetta cortina di ferro, aveva condannato questi nostri fratelli europei ad un periodo buio e difficile da superare. Ma oggi la realtà dei Paesi dell'Europa dell'Est, pur comprensibile per le ragioni ed i motivi di carattere politico, storico e culturale, rappresenta un'anomalia all'interno dell'Europa. Non è un caso - credo si debba prenderne atto che vi è più un avvicinamento all'Europa in quanto NATO, in quanto sicurezza, garanzia da parte degli Stati Uniti d'America che non un approccio all'Europa in quanto Europa, in quanto possibilità o capacità di ricevere dall'Europa quegli aiuti che evidentemente questi si aspettano. Credo vi sia un po' anche la sindrome dell'accerchiamento. Si usa dire, con una battuta forse cattiva, che quando la Russia è grande la Polonia è russa, quando la Germania è potente la Polonia è tedesca e quando i due sono molto deboli la Polonia è libera. Questa è la storia millenaria della Polonia. Noi ci inchiniamo anche alla storia polacca, ma evidentemente in questo momento il peso della storia ha influito negativamente sul processo europeo, così come influiscono negativamente l'accordo sullo scudo spaziale, sullo scudo spaziale, o l'appoggio o le posizioni assunte su materie come l'ingresso della Turchia in Europa. Allora prendiamo atto anche di questo aspetto. Prendiamo atto di una volontà britannica. Chissà, forse aveva ragione il generale De Gaulle, che non aveva mai considerato l'Inghilterra una quota di appartenenza all'Europa. Forse aveva ragione chi, con una battuta che ho trovato molto felice, ai tempi della guerra irachena pensava che Blair ritenesse di essere ancora a capo dell'Impero e che gli americani fossero ancora la colonia che ubbidiva agli ordini di Londra. Anche questa è una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, ma noi vogliamo andare avanti sulla strada dell'Europa.

Alla fine si dice: «a collocare, comunque, in ogni futuro sviluppo del negoziato, il nostro Paese nel nucleo di avanguardia di una più stretta integrazione, anche facendo ricorso allo strumento istituzionale delle cooperazioni rafforzate». Io non posso non essere d'accordo, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, basta che ci intendiamo con grande serenità e senso della realtà, su una questione: stiamo auspicando un'Europa a doppia velocità. Stiamo auspicando che alcuni grandi Paesi europei, non solo i fondatori (penso alla Spagna, che si potrebbe unire a questo nucleo forte e duro o forse ai Paesi che hanno accettato l'euro), si facciano promotori di una politica più forte, certamente attraverso lo strumento delle cooperazioni rafforzate, ma non come fatto tattico, argomento per argomento, bensì come strategia complessiva che individua alcune materie fondamentali (perché non pensare alla politica estera o alla politica di difesa?), sulle quali tali cooperazioni rafforzate possano indicare un'Europa che continua secondo i tempi auspicati prima di Bruxelles. Su questa strada dell'Europa a due velocità mi ricordo anche le dichiarazioni del presidente Prodi, al quale peraltro devo dire con grande onestà intellettuale che ci aspettavamo di più dalla posizione italiana, dopo le sue dichiarazioni, non le nostre, che erano state fatte prima dell'incontro di Bruxelles, ma io dico oggi con un certo coraggio, forse considerando anche che il multilateralismo è uno strumento della politica estera, e che nel caso delle cooperazioni rafforzate ritorna il valore dei rapporti bilaterali tra i Paesi europei, quindi il valore di una politica bilaterale che costruisce una politica multilaterale, non il contrario. Su questo credo si possa tutti assieme ritrovare quell'unità di intenti che le forze politiche presenti in questo Parlamento avevano trovato nella primitiva risoluzione Manzella. Questo è l'auspicio. Non penso si debba debba esprimere nessun giudizio o critica su quanto avvenuto a Bruxelles. Occorre con grande serenità e realismo politico prendere atto di questa Europa, che probabilmente è un grande Commonwealth di regole, di procedure, di interessi importanti, di sviluppo economico, di moneta unica, che però non è priva di anima: è priva di politica, di grandi obiettivi strategici. Credo che il compito dell'Italia ritorni ad essere quello degli anni Cinquanta: tornare a essere protagonista, insieme agli altri Paesi, di un rilancio di questa Europa, pensando all'Europa a 27, che poi si allargherà ancora. Penso con grande preoccupazione - devo dire - ad un'Europa che si allarga ai Paesi dei Balcani., penso con grande preoccupazione ad un Kosovo indipendente, come molti auspicano e vogliono, contrariamente ad ogni logica della politica. Forse questa Europa troppo allargata e ricca di problemi - i Balcani ce ne porteranno molti - non ha bisogno di molti

che, pur non avendo firmato e non firmando la proposta di risoluzione, preannuncio che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore della

dei tempi contingentati. Condivido anche la scelta di limitare la discussione di oggi ai principali temi, che sono stati affrontati così bene da quest'Assemblea stamattina,

ulteriore lento ma inesorabile declino di un'Europa alla quale guardiamo spesso con fiducia, che viene disattesa e delusa, come ha raccontato molto bene prima il senatore Mantica, nella quale però noi continuiamo a a nutrire una fiducia incrollabile. Sappiamo che in passato il cammino di questa Europa è stato anche più difficile di questo. Tuttavia, grandi uomini e Governi lungimiranti non hanno mai perso la speranza di costruire il sistema dentro il quale oggi tentiamo di svolgere un ruolo che da tanto tempo non svolgiamo più. Aveva perfettamente ragione, senatore Mantica, quando prima rimpiangeva e ricordava lo spirito di partecipazione dei Governi dell'epoca, negli anni Cinquanta, che hanno fatto grande, grandissima l'Europa di quel tempo, mettendo in moto un meccanismo di unione economica, innanzitutto, che si è concluso nella

nelle procedure e nelle modalità, presidente Manzella, che pure faticosamente tentiamo di conciliare con il nostro entusiasmo

d'intendere e di organizzare la discussione sulla legge comunitaria è sbagliato. Forse oggi possiamo compiere un ulteriore passo in avanti su questo processo faticoso e su questo cammino così difficile. Abbiamo l'obbligo di interrogarci se il nostro modo di affrontare il tema della legge comunitaria è esattamente corretto o se non valga la pena, come molti

questa possa essere una delle ultime leggi comunitarie che recepiamo in questo modo poco intelligente, poco efficace poco efficace e direi anche poco democratico e rispettoso per i cittadini e le genti che dovremmo rappresentare. Noi nel recepimento della legge comunitaria non rappresentiamo solo le istanze degli italiani, ma partecipiamo a un processo, e tutta la nostra lacuna di rappresentanza, dal punto di vista politico oltre che da quello civile, emerge in questa fase. Sappiamo esattamente cosa cosa serve ai cittadini italiani all'interno dell'Europa e quindi cosa serve all'Europa? Penso di no e penso che dovremmo riuscire a fare uno sforzo oltre i confini della politica estera, che è parte fondamentale e fondante dell'Unione Europea, nel comprendere meglio alcuni meccanismi di natura economica che incidono pesantemente e pesantemente condizionano il giudizio di tanti cittadini, di tanti popoli che pure formalmente appartengono all'Europa, ma che quell'Europa non sentono vicina. Anche in questa nostra procedura c'è infatti l'evidente dimostrazione che siamo ancora all'Europa delle burocrazie e che siamo di fronte ad un'Europa senz'anima, che non riusciamo a riempire di contenuti e di anima. e molte altre ancore che il senatore Stiffoni ha segnalato questa mattina. Sappiamo bene che c'è una legge che ci impone di fare questo, ma forse è il momento di rivederla e di confrontarci su quale sia il modo migliore per rendere fruibile e vera questa Europa riempirla di anima e di contenuti, anche attraverso le sue procedure e le sue forme. Quindi le mie due proposte fondamentalmente riguardano come viviamo questo processo e come questo Parlamento lo può rendere più efficace e democratico possibile. La modalità prevista dalla legge Buttiglione probabilmente va riformata e modificata; spero che tutti noi, a prescindere dai nostri schieramenti, come sempre facciamo in occasione dei grandi appuntamenti europei, avremo la forza, la capacità e l'onestà intellettuale di migliorare questo percorso. Così, questo Parlamento dovrebbe potersi occupare nella sua totalità di questioni assai rilevanti, che spesso pochi conoscono e che non aiutano il processo di crescita e di sviluppo della testa politica - che prima di essere politica è culturale dell'Europa, che invochiamo e che puntualmente vediamo latitante. Ci troviamo infatti di fronte ad un'Europa fatta di gambe senza testa, che comunque continuano a procedere e a camminare in una direzione alla cui decisione alla cui decisione spesso non partecipiamo. Dunque, contro questa Europa che rischia di finire sotto l'egemonia totale delle burocrazie dobbiamo saper invocare gli strumenti della politica nel rispetto della democrazia e soprattutto,

l'ho presentata per capire se il Vice ministro ancora eserciti la delega sulla Guardia di finanza. La questione è stata sollevata in Aula anche dal presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Matteoli, nonché dal senatore Eufemi. argomento non abbiamo avuto nessuna risposta da una decina di giorni, ma i solerti uffici del mio Gruppo hanno trovato invece un decreto ministeriale - si noti bene: un decreto ministeriale - del vice ministro Visco datato 1° giugno